recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)

Signor Presidente, colleghe e colleghi, dall'inizio della legislatura credo non ci sia stato ancora un provvedimento importante trattato dai due rami del Parlamento, quindi anche questa volta devo cominciare il mio intervento denunciando quest'anomalia, che tale resterà fino a quando non si metterà mano al bicameralismo perfetto. Tuttavia, almeno in questo caso, con un po' di fortuna e di collaborazione, possiamo dire che il Senato ha avuto un ruolo nel determinare l'indirizzo del provvedimento con gli ordini del giorno impegnativi approvati nel primo quindi, di un provvedimento positivo, non solo per la mole delle risorse, ma anche perché risponde puntualmente a una serie di questioni. Penso anzitutto agli interventi a copertura dei costi fissi delle imprese, sui rifiuti (TARI), a quelli sul credito d'imposta, alle misure per favorire l'accesso al credito e scongiurare crisi di liquidità. Penso alle misure di sostegno per il mondo del lavoro, col rifinanziamento della NASPI e di ulteriori mesi di cassa integrazione, di aiuti a fondo perduto per i lavoratori autonomi. Penso naturalmente all'incremento del Fondo nazionale per la montagna, per sostenere le attività capofiliera, i maestri di sci, le imprese e l'economia della neve, che (non dimentichiamolo) è stata quella più colpita dalle restrizioni della seconda ondata. Un altro elemento importante per la montagna introdotto col primo decreto-legge ristori è stata la scelta del periodo di riferimento per il calcolo dell'indennizzo. Come ha ricordato in audizione il ministro Franco, i numeri ci hanno dato ragione e le imprese che hanno optato per il calcolo sull'anno pandemico ottengono indennizzi più congrui. Presidente, se queste sono le tante note positive, bisogna fare uno sforzo ancora più grande sui decreti attuativi per l'erogazione fattiva delle risorse. Solo con questo provvedimento ne sono necessari 41, che si vanno ad aggiungere ai 28 del primo un imbuto burocratico che sta facendo montare la preoccupazione tra gli operatori del turismo invernale, visto che gli aiuti arriveranno non prima di settembre per gli impianti di risalita e non prima di ottobre per le scuole e i maestri di sci. So perfettamente che siamo in una situazione eccezionale, che è davvero grande lo sforzo che stiamo facendo, ma dobbiamo capire che è nulla rispetto allo sforzo che stanno facendo numerose imprese nel non gettare la spugna. Dobbiamo anche capire che non ci sarebbe sciagura più grande di una nuova stagione di restrizioni e di chiusure. La scienza ce lo dice chiaramente: se è vero che sono diminuite le ospedalizzazioni, più il *virus* gira, più aumenta il rischio di una variante in grado di bucare il vaccino. Quindi massima attenzione, massima prudenza, ma soprattutto programmare la gestione dell'autunno attraverso i tracciamenti e una maggiore centralità del *green pass,* del *green pass,* che non è una minaccia alla libertà individuale, ma uno strumento transitorio per incentivare le vaccinazioni ed è anche una forma premiale per tutti quelli che, vaccinandosi, hanno compiuto un gesto utile non solo per sé, ma per l'intera collettività. caso so che non è una scelta semplice, che il Paese vorrebbe lasciarsi finalmente alle spalle la pandemia, ma se non facciamo adesso un passo in avanti, rischiamo di farne diversi indietro nel giro di poche settimane. Presidente, il provvedimento in discussione pesa 40 miliardi, un'altra massiccia iniezione di risorse per le famiglie e le imprese, che però non basteranno se non si consoliderà il duplice impegno contro la pandemia e per lo sviluppo del PNRR. Ne riparleremo quando arriverà il decreto-legge sulla *governance,* in particolare sul ruolo che devono avere gli enti locali superando le problematiche che stanno emergendo sulle autonomie speciali. però, vale lo stesso ragionamento sul *green pass:* le decisioni non sono facili, ma mai come in questa fase storica occorre decidere sempre in termini di interesse generale. Spero quindi davvero che non si smarrisca quello spirito di unità nazionale sollecitato dal presidente Mattarella al momento della nascita di questo Governo. Quel principio non può valere solo quando si tratta di fare politiche redistributive, ma anche quando si devono sviluppare tutte le condizioni per attuare il PNRR, dalla riforma della giustizia, a quella del fisco, dall'obiettivo dell'immunità di gregge, alle altre misure per evitare nuove restrizioni e chiusure. La corsa a differenziarsi, a sopire, ad annacquare, a mettere le mani avanti oggi non aiuta né il Paese né le stesse forze politiche che lo fanno. Gli italiani sanno che questa fase richiede scelte robuste e coraggiose, scelte che dobbiamo sostenere con maggiore convinzione, anche esponendoci a qualche rischio di impopolarità, perché è chiaro che ci sarà sempre una parte a cui certe decisioni non vanno bene. Noi come autonomisti ci siamo sempre stati e continueremo ad esserci ed è per questo che annuncio il voto favorevole del Gruppo al provvedimento e rinnoviamo la fiducia al Governo.

per farle presente che in tutta questa legislatura e, in particolare, dalla dichiarazione dello stato d'emergenza, il rapporto tra legislativo ed esecutivo è stato critico e che il ruolo del Parlamento è stato particolarmente compresso. sostegni-*bis* è un provvedimento necessario e importante, che impegna quasi 40 miliardi di risorse. È altresì un provvedimento che noi abbiamo fortemente indirizzato perché ricordo un ordine del giorno predisposto dalla Commissione bilancio a chiusura e ad approvazione del sostegni-*bis*

Nel merito è un provvedimento buono e tecnicamente fatto bene, che supera anche tre criticità che in tutto l'anno pandemico ho evidenziato come particolarmente pericolose, non solo per la nostra economia, ma anche per il nostro Stato di diritto. Penso al superamento degli interventi a pioggia con stampo assistenziale. La nuova impostazione dei contributi a fondo perduto, che pure deve chiudersi con questo ultimo è stata molto più mirata e focalizzata sul calo del fatturato e sulle effettive necessità delle imprese. Penso al superamento del blocco degli sfratti, una misura fortemente critica per il valore e il principio costituzionale della proprietà privata. È stato finalmente parzialmente sbloccato e sono state anche pensate misure per indennizzare i proprietari di immobili con l'esenzione IMU per chi avesse una convalida di sfratto e per la dichiarazione di non tassazione

del blocco dei licenziamenti; sappiamo che è stata una mediazione piuttosto faticosa, che era però assolutamente necessaria. L'Italia è stata tra i pochissimi Paesi al mondo ad adottare questo tipo di impostazione e di misura, peraltro grandi risultati perché i numeri della disoccupazione sono pari a quelli di altri Paesi europei ed è stata l'ultima a rivederla. Siamo quindi assolutamente favorevoli misura. Complessivamente il mio giudizio sul provvedimento è positivo e quindi la mia critica riguarda il metodo di approvazione più che il merito. Ormai siamo a un monocameralismo alternato; siamo in uno stato in cui le Commissioni lavorano avendo pochissimo tempo per analizzare i provvedimenti. con il lavoro di collaborazione tra i Gruppi parlamentari di Camera e Senato può decidere di fare emendamenti alternati, mettendosi politicamente d'accordo sulle priorità, certamente il lavoro Parlamento e del legislatore non può essere compresso nella possibilità di studio e di approfondimento dei provvedimenti. Affermo inoltre con chiarezza che nemmeno la possibilità di indirizzo politico può essere compressa da scelte tecniche delle amministrazioni che, in realtà,

che fosse il momento che le istituzioni avessero un assetto più efficiente; eppure, gli italiani hanno detto no, hanno detto che si fidano della doppia lettura, quindi non solo di deputati e senatori, ma si fidano dei tecnici di Camera e Senato. Questo mandato dobbiamo rispettarlo. dobbiamo rispettarlo. Il mese di luglio nella nostra impostazione parlamentare deve segnare uno iato, una divisione di tempi. Finiamo l'epoca pandemica; sappiamo che i vaccini usati sapientemente sapranno riportarci alle nostre attività in sicurezza, e sappiamo anche che dal 13 luglio abbiamo il via libera - della Commissione, prima, e dell'Ecofin dopo - al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Abbiamo cinque anni nei quali trasformare l'Italia: dall'alta velocità all'intermodalità, dall'intelligenza artificiale all'economia sostenibile. Abbiamo da fare un lavoro straordinario. Non tutti i cinque anni competono a noi;

Parlo delle riforme di accompagnamento, delle riforme orizzontali al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Presidente, quelle riforme non possono essere affrontate con un monocameralismo; c'è bisogno di una forte collaborazione, di una forte messa a sistema del Governo, sicuramente con l'Europa - e questa certamente c'è - ma anche con il Parlamento.

che se l'Italia non vince la sfida del Piano nazionale di ripresa e resilienza non resterà nel G7. Ci sono dei previsori - magari non amanti dell'Italia

di Italia Viva vogliamo un'Italia che resti nel G7 e vogliamo una parola, che forse è brutta e si pronuncia SAL: un acronimo decisamente cacofonico, significa stato avanzamento lavori. Questo è l'unico acronimo che deve rimbalzarci nella testa ogni giorno dei prossimi cinque anni. Presidente, i 240 miliardi ad oggi sono nominali; arriveranno solo se questo Parlamento e il Governo - questo e il prossimo - saranno capaci di fare

è necessario perché è prodromico alla ripartenza, l'unica cosa che in questo momento realmente conta assieme alla capacità di trasformare l'Italia. Sosteniamo il Governo con grande convinzione e lo ringraziamo per il lavoro di alta qualità che ogni giorno svolge per l'Italia e per gli italiani. [DE

provvedimento e spiego perché siamo contrari sia nel metodo che nel merito. Nel metodo perché è ormai palese - lo dicono anche i colleghi che mi hanno preceduto, come se fosse colpa di qualcun altro, non degli stessi il ricorso compulsivo alla decretazione d'urgenza, anche se la pandemia ormai non è più un'urgenza. Dopo un anno e mezzo di confronto costante e continuo con questo disagio che ha colpito la Nazione e il mondo, pensare che qualcosa sia urgente ed emergenziale significa sancire il fallimento della politica di programmazione e della visione dei vari Governi che si sono succeduti all'unico scopo, stante le vostre dichiarazioni, di salvare questa Nazione. Ripeto, salvare da chi, poi, se non da coloro che avevano contribuito a farla arrivare sul baratro? Quelli che oggi fanno parte del Governo Draghi sono gli stessi che - guarda caso - facevano parte dei Governi precedenti, quindi è un'altra ammissione di fallimento rispetto solo a qualche mese prima.

i parlamentari salivano sui tetti di Montecitorio per manifestare la loro contrarietà alla fiducia e lo facevano giustamente, credendo che si privasse chi era democraticamente eletto come membro del Parlamento della possibilità di incidere sui provvedimenti. Ebbene, oggi quegli stessi parlamentari sono quelli che abbassano gli occhi e trovano una giustificazione - chi richiamando l'emergenza, chi il fatto di dover salvare la Nazione - a questo

la maggior parte di voi ha votato sicuramente no, come tanti cittadini, al *referendum* del 2016 sull'abolizione del Senato. Oggi invece tradite quel mandato dei cittadini con un ricorso alla fiducia che di fatto sancisce il costante e continuo monocameralismo, cioè la possibilità per noi di discutere un provvedimento in una Camera sola, come se l'altra non servisse, come se il mandato popolare che c'è stato dato da milioni di cittadini non servisse a nulla. Oggi infatti c'è questa grande "macedonia" di Governo - guarda caso sempre con una logica di accordo al ribasso che salva la Nazione e quindi non c'è nemmeno bisogno di quello spicchio di deputati e senatori di Fratelli d'Italia che quasi sono percepiti come un ingombro,

tendete a discriminare e perseguitare chi ha una visione differente dalla vostra e dedicate appunto a quel provvedimento molta più discussione di quella che dedichiamo ad un provvedimento da 40 miliardi che dovrebbe risolvere o proverebbe a risolvere i problemi di tante imprese. Il disegno di legge Zan probabilmente sposterete a settembre, quando più vi servirà in campagna elettorale, quando qualcuno di voi lo agiterà come una bandiera a tutela della libertà. Noi invece la bandiera a tutela della libertà la sventoliamo tutti i giorni, anche solo con la nostra presenza in Aula. Non esiste un Paese al mondo che si dica o che sia democratico in cui non esiste l'opposizione, fatevene una ragione, e quell'opposizione è rappresentata proprio da noi, che quindi ci permettiamo anche di dire cose che magari a voi sono un po' scomode. La democrazia si pratica, non si predica, questo è un concetto fondamentale, non potete insegnare la democrazia quando praticate l'antidemocrazia e scambiate l'autorevolezza che credete di avere con il vostro autoritarismo. Capisco che per molti di voi questo sia fonte di assoluta vergogna, dopo aver passato la vita a sbandierare la democrazia come un valore insito nel vostro DNA. Purtroppo poi alla prova dei fatti vi siete dimostrati quello che in realtà siete: liberticidi, limitatori delle libertà altrui, altrui, coercitivi della libertà dei cittadini. Io ho avuto il Covid, mi sono vaccinato come tanti di noi, ma credo che non possiamo obbligare qualcuno a farlo solo per il nostro desiderio

AstraZeneca sì, AstraZeneca no, la copertura delle varianti sì, la copertura delle varianti no - avete determinato l'incertezza in tanti cittadini italiani che oggi non si stanno vaccinando. è la base scientifica? Qualcuno in questa Aula può alzarsi e dire che oggi può certificare con assoluta certezza che chi è vaccinato non è in grado di contagiare? Mi pongo un'altra domanda: perché la stessa ferma volontà sui vaccini non la mettiamo in campo anche quando si tratta di curare questo virus? Ci siamo ormai convinti che non c'è rimedio a questo virus, che non esiste possibilità di cura, che l'unica cosa cui dovremmo abituarci è una dose mensile, semestrale o annuale di vaccino? Qualcuno me lo sa dire? sa dire? In un'Aula di tuttologi come questa, c'è qualcuno che può scientificamente rispondere a queste domande? Se ci fosse, non farebbe chiarezza solo a me che sono vaccinato, ma anche a quelli che fino ad oggi non hanno deciso di farlo proprio per la confusione che voi avete generato nei cittadini. E non voglio nemmeno credere che lo facciate per mantenere uno stato di emergenza perenne che vi consente di calpestare ogni forma di democrazia qui dentro e fuori da queste istituzioni. Se non ci fosse lo stato di emergenza oggi, voi non esistereste nemmeno. Saremmo già andati a votare tutti, come votano milioni di cittadini nelle città più importanti d'Italia. Gli unici per cui non si vota siamo noi perché avete paura di andare a casa; avete paura del giudizio popolare e non perché l'opposizione stia facendo falsa o distorta informazione. Basta la vostra confusione! Il cittadino è molto più maturo di tanti di voi; il cittadino non deve preservare la propria poltrona. Il cittadino fuori giudica in base a ciò che vede; e vede una maggioranza raffazzonata che segue sempre la logica del ribasso e che fa di tutto per rimanere in quest'Aula abbarbicata alla sua poltrona.

Poco vi interessa se uno su quattro non sarà in grado di andare al ristorante, se mettete il certificato obbligatorio. Non vi interessa nulla; non vi interessa se qualcuno non può avere il *green pass* perché ha delle malattie e non può vaccinarsi. Non vi interessa. Vi importa solo far passare il vostro messaggio liberticida per cui uno si comporta come volete voi o è un dannato. Signori, non è così. Voi dovete fornire gli strumenti scientifici a supporto delle vostre tesi, altrimenti siete dei *guru* del nulla e non si legifera in una Nazione con il nulla, ma con la scientificità degli atti. Ciò vale solo per il metodo. Nel merito non dovrei neanche intervenire. Dovrei stendere un velo pietoso.

non per deliberare sul nulla, per avere uno *slogan* e fare un *tweet*, per rincorrervi su chi è il più bravo. Risorse non se ne vedono. Le imprese ci chiedono ben altro.

sarebbe potuto servire ad abbassare il costo del lavoro delle imprese. È inutile, infatti, dirsi contro i licenziamenti se poi non si danno gli strumenti a quelle imprese per lavorare. Il provvedimento è pessimo e in assoluta continuità con i provvedimenti che abbiamo sempre visto con il Conte I, II e con il Governo Draghi. Pertanto, non avrete mai la nostra fiducia. Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, accompagnare il Paese fuori dalla crisi e, al tempo stesso, scongiurare danni permanenti al nostro tessuto produttivo, insieme al consolidamento della ripresa in atto, anche per aiutare, sostenere e favorire l'uscita dalla crisi e la ripartenza della nostra economia, sono i cardini fondamentali del decreto sostegni Essi rappresentano, per il nostro Paese, non solo in termini quantitativi, ma anche per la scelta politica e culturale che sta alla base di questi decreti, le radici fondamentali dell'identità del Paese. I 76 miliardi di euro sono utilizzati per sostenere le imprese, per aiutare le partite IVA colpite dalle difficoltà della pandemia, per sostenere il sistema sanitario pubblico nell'attraversare una fase molto difficile e complessa della vita economica e sociale del nostro Paese. In quanta difficoltà si è consolidato quel diritto alla salute, che le risorse che abbiamo destinato hanno aiutato a consolidare! I capisaldi di questi decreti-legge sono le ragioni fondamentali per le quali esprimiamo non solo la conferma della fiducia nei confronti del Governo, ma anche una condivisione di metodo e di merito, sulla quale abbiamo consolidato le azioni fondamentali, che hanno portato l'identità del Partito Democratico ad attraversare questa fase di crisi pandemica, attraverso principi e valori molto importanti, che non dobbiamo mai dimenticare: il sostegno al lavoro, ma nello stesso tempo la consapevolezza che c'era un ritardo culturale da colmare nel sostegno e nella protezione di una moltitudine di partite IVA, di piccole e medie attività,

alla qualità della vita dei nostri centri storici e della nostra economia. È stato dunque un lavoro fondamentale, che aveva radice nel non lasciare da sole le persone e nel non lasciare da sole le imprese. Non c'è conflitto possibile tra capitale e lavoro dentro queste dinamiche. C'era l'obiettivo di unire il Paese, in un grande sacrificio complesso e difficile, per uscire da questa crisi pandemica. Diciamo francamente che abbiamo utilizzato 200 miliardi di euro di indebitamento netto nel 2020 e 76 miliardi abbiamo portato il rapporto tra *deficit* e PIL all'11,8 per cento e, se a questo aggiungiamo le fondamentali e importanti risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, due terzi delle quali anch'esse ad indebitamento netto, siamo di fronte ad un obiettivo cruciale: essere consapevoli che la sostenibilità del nostro debito passa attraverso una nuova crescita strutturale e attraverso la rimozione di quei problemi strutturali che l'Italia ha sempre avuto, nella bassa crescita. Lo dico perché le riforme che accompagnano questi provvedimenti sono fondamentali per affrontare temi strutturali, che tenevano l'Italia tra i Paesi con la più bassa crescita economica nella dimensione europea. Pensate al tema dei giovani, dell'altissimo tasso di disoccupazione giovanile, pensate ai temi della natalità, perché oggi il tema fondamentale sarà proprio quello di mettere a disposizione del Paese e di questa nuova crescita economica le risorse umane sufficienti per abbracciare il futuro. La conversione in chiave ecologica dell'economia e la transizione ambientale e digitale, ma allo stesso tempo anche la transizione sociale, che dobbiamo costruire e programmare, richiedono uno sforzo nuovo sul versante della formazione e della promozione delle competenze. Già oggi non siamo abituati ad una crescita del 6 per cento, perché pur di fronte ad una caduta del PIL del 9

mettiamo al centro i processi della formazione e dell'istruzione, perché non c'è futuro se non accompagniamo una conversione delle risorse umane indirizzate ad essere protagoniste di questa nuova crescita. Siamo condannati a crescere strutturalmente oltre 2 punti e mezzo di PIL, per rendere sostenibile il nostro debito. È dunque evidente - e lo dico con grande franchezza - che ci sentiamo orgogliosi anche del lavoro svolto nel precedente Governo, e ancora rafforzato da questo Governo, nella costruzione del nuovo volto dell'Europa. Next generation EU compie un anno; sembra un secolo, ma in realtà è un anno che abbiamo di fronte un nuovo volto dell'Europa: un'Europa che si appresterà, attraverso il Next generation EU, a rendere strutturale una riforma del Patto di stabilità, perché si cancellerà finalmente l'Europa dei "segni meno", dei tagli lineari, dell'*austerity*, dell'esclusiva attenzione alla dimensione economica. Ci sarà infatti inevitabilmente bisogno di di rendere strutturale Next generation EU per favorire strutturalmente una crescita più alta. È evidente che l'utilizzo veloce delle risorse e, nello stesso tempo, l'indirizzo delle risorse verso la transizione vanno perseguiti con coraggio e senza ambiguità: infatti costare di più una manutenzione ordinaria dell'esistente che un investimento che occupi e promuova nuova economia. Dobbiamo prendere in mano le filiere produttive; dobbiamo costruire un piano regolatore dello sviluppo economico. Ci vuole un piano regolatore, perché l'Italia deve inevitabilmente scegliere quali sono le direttrici fondamentali del proprio sviluppo economico. Se coglieremo questa opportunità, un nuovo volto dell'Europa, caratterizzato dalla riforma del Patto di stabilità, dal consolidamento di Next generation EU, da una riforma orientata verso la sostenibilità economica, da una nuova crescita economica, dalla transizione energetica, digitale e sociale. Il Patto di stabilità dovrà favorire gli investimenti, non bloccarli, come è successo prima della pandemia. Ci sentiamo figli di questo nuovo europeismo: il Partito Democratico ha lì le sue radici.

Il protagonismo dell'Italia nei confronti dell'Unione europea è indispensabile per consolidare questo progetto. Non c'è spazio per abbracciare Orbán strutturalmente e politicamente, per una foto o un messaggio ambiguo. Non c'è spazio nemmeno per correggere i limiti che ci possono essere stati nella comunicazione, nell'esercizio delle funzioni e anche nella promozione delle campagne vaccinali. Nessuno nega che ci sono stati limiti, ma per noi - lo dico chiaramente - non si correggono questi limiti rinunciando alla scienza, rifiutando o contrastando le indicazioni della comunità scientifica. *(Applausi)*. Anzi, si crea un danno micidiale:

Un insegnante, al pari di un medico, rappresenta un pezzo fondamentale dell' articolazione dello Stato; è il responsabile di una comunità educativa.

per quello che è stato il lavoro della Scienza, è indispensabile per proteggere non solo l'individuo singolo, ma soprattutto la comunità dentro la quale abita. Le mie libertà iniziano quando anche chi abita vicino a me è libero di potersi muovere, costruire e progettare il proprio futuro. Non ci vogliono ambiguità. Lavoriamo dunque

della campagna vaccinale, perché questo è indispensabile per consolidare l'uscita da questa crisi. Facciamolo insieme, senza ambiguità e abbracciamo finalmente quel processo del nuovo europeismo che renderà l'economia e la società italiane più giuste, più eque e più solidali.

è frutto anche del lavoro fatto dal Senato, come alcuni colleghi hanno già evidenziato. Con gli ordini del giorno

di segnali utili. Vedo che continua una polemica francamente un po' riguardante le grandi novità del Governo Draghi rispetto al Governo Conte. Voglio ricordare a tutti i colleghi che

modo, è stata fondamentale la capacità, anche con il reddito di emergenza, di rispondere ai buchi esistenti. Questo non significa che sul reddito di cittadinanza non vi sia la necessità di fare degli interventi correttivi. Ma è una scelta che hanno fatto praticamente tutti i Paesi europei; io vorrei che ne prendessimo atto e che riuscissimo a fare un salto di qualità nella discussione.

C'è una grande questione salariale nel nostro Paese; senza affrontare questa, non andiamo da nessuna parte.

È un intervento *spot* che non risolve il problema. C'è un ordine del giorno che il Governo ha approvato, presentato da noi, che sollecita a impostare una nuova politica del farmaco, una nuova *governance*. È giusto rivedere i tetti, ciò va fatto all'interno di una strategia di sistema; diversamente, il sistema sanitario non reggerà. Colleghe e colleghi, i nuovi farmaci innovativi hanno dei costi

C'è già un documento sulla *governance*, è dentro al Patto per la salute: applichiamolo subito e rivediamo il prontuario farmaceutico, dove paghiamo dei farmaci il 150 o il 200 per cento in più di quello che si dovrebbero pagare. Bisogna fare delle scelte, e arrivo così all'ultimo punto che volevo sollevare. La discussione è stata complessa. Capisco bene che siamo in una situazione difficile e che non si può recriminare

si possono anche convertire i decreti-legge in poco tempo, ma lo spazio per un confronto politico ci deve essere. Prima di impostare il provvedimento e durante l'impostazione del provvedimento, il Governo ci faccia una proposta; non possiamo trovarci costretti in un monocameralismo di fatto, che ci impedisce di dare un contributo. È un compito fondamentale del Governo quello di valorizzare il ruolo e i contributi che vengono dai Gruppi parlamentari. Valorizzare quest'Aula non è un elemento di debolezza, ma è un elemento di forza del Governo. A questo proposito, vorrei dare alcune indicazioni di lavoro. Al di là dei decreti - su cui pure bisognerà trovare con il Ministro per i rapporti con il Parlamento un percorso diverso - vogliamo discutere della direzione di marcia del PNRR? È ora. Io sono preoccupato quando sento Ministri che ci dicono che la proposta della Commissione europea sulla transizione ecologica è troppo rapida. Quale strada stiamo prendendo? Che riforma del *welfare* stiamo attuando? Come vanno i progetti? Per valorizzare l'Aula, non serve stabilire che c'è una quota che si distribuisce tra i diversi Gruppi. A me di questo non interessa nulla.

fra qualche mese, al primo *check* sui progetti, a verificare che siamo in ritardo e magari incrociare a quel punto progetti già fatti,

Io dico che dobbiamo lavorare perché dopo la pandemia cambi davvero questo Paese.

come già detto da numerosi colleghi prima del mio intervento, anche oggi votiamo in quest'Aula un provvedimento cristallizzato in un in un solo ramo del Parlamento: una prassi che potrebbe anche avere le sue motivazioni, ma che certo non rispetta oggi il dettato costituzionale, che prevede l'attività legislativa in capo alle due

importante, che nasce con una base di 40 miliardi e 77 articoli; poi, nel lavoro parlamentare che è stato fatto alla Camera, si reperiscono altre risorse

Siamo in emergenza, dobbiamo essere veloci nelle misure. *(Applausi)*. Quindi, Sottosegretario, invito lei e il Governo a dare attuazione immediata a tutti i decreti attuativi che ci sono, perché bisogna arrivare

dal Parlamento, come scostamento di bilancio: una vera e propria manovra finanziaria. Le modifiche alla Camera hanno assolutamente migliorato il provvedimento, lo hanno potenziato, soprattutto sulle misure economiche, che oggi devono avere un forte impatto sociale ed economico, perché sappiamo tutti come la pandemia ha portato quest'anno a una grave crisi. Una Una ripartenza che - sappiamo tutti - non è facile; ce lo dicono i dati economici, ce lo dice anche l'Istat: ci sono interi comparti industriali che stentano ancora a ripartire. Abbiamo quindi la necessità di aiutare e sostenere

che scontentavano tutti, così come abbiamo eliminato tante forme di assistenzialismo che non servivano a niente e siamo passati al fondo perduto, agli investimenti: tutte linee di indirizzo che Forza Italia ha dettato nei vari provvedimenti.

poi anche l'accesso al credito e alla liquidità per le imprese: 9 miliardi di euro per garantire l'accesso al credito, sostenere la liquidità e incentivare la capitalizzazione. È stata prorogata al 31 dicembre 2021 la moratoria sui prestiti. Si tratta quindi di tanti provvedimenti importanti

è stato l'impatto devastante della pandemia sul sistema economico italiano, che è fatto di piccole e medie imprese, che non possono resistere tanto in autonomia. Ecco dunque perché il sostegno, il supporto alle attività economiche, che non abbiamo fatto mancare. un colloquio diretto con le categorie produttive, con i professionisti, con le partite IVA. Li abbiamo sempre ascoltati; abbiamo preso e acquisito le loro proposte e le abbiamo trasformate in provvedimenti, perché abbiamo un collegamento diretto con le imprese.

a preparare tutti quei provvedimenti che oggi anticipino l'emergenza che può determinarsi. È importante essere pronti. Ecco perché non dobbiamo mollare, ma essere tempestivi e incisivi,

Per noi rappresenta un vero e proprio cambio di passo e di impostazione rispetto ai decreti-legge ristori del precedente Governo. Innanzitutto non ci sono sprechi, né scelte discutibili. Tutta l'opposizione ha mosso legittimamente critiche al metodo, ossia al fatto che questa Camera non abbia potuto emendare il provvedimento; sicuramente di critiche importanti, ma non una critica è stata mossa rispetto alle norme contenute in questo decreto-legge, a dimostrazione che c'è stato un cambio di passo e non sono stati stanziati fondi in direzioni discutibili, come avvenuto in passato per monopattini, banchi a rotelle, *bonus*, sussidi. *(Applausi)*. Questo rappresenta un cambiamento di cui la Lega si è resa protagonista. Ogni misura è stata indirizzata al sostegno di chi ha subito i danni più pesanti della pandemia e al rilancio della nostra economia. Sono poi cambiati i criteri: rispetto ai decreti ristori del Governo Conte, non si sono più utilizzati i codici Ateco - alcuni sì e alcuni no - per erogare i sostegni. Finalmente ci si è basati sul calo del fatturato, come è stato richiesto a più riprese dalla Lega quando era all'opposizione, ed è stato utilizzato come criterio la perdita dei costi fissi d'esercizio. Questo è il contributo che la Lega ha dato a questo provvedimento e al cambio di passo di questo Governo. a differenza dei decreti-legge ristori del Governo precedente, il provvedimento aiuta i dimenticati. Sono stati garantiti sostegni partite IVA, autonomi e al settore del turismo (hotel, ristoranti, bar), al settore del *wedding*, alle fiere nazionali, ai centri termali, agli impianti di risalita sciistici, alle agenzie di viaggio, ai bus turistici, alle guide turistiche: tutti settori che nei precedenti decreti erano stati tralasciati e trascurati. Non abbiamo dimenticato il terzo settore, l'IPAB la non autosufficienza e nemmeno gli agricoltori, colpiti da gelate, alluvioni e calamità naturali. Abbiamo finalmente stabilito un criterio di giustizia nei confronti dei proprietari degli immobili affittati. Abbiamo tutelato chi ha subito il blocco degli sfratti, che non dovrà pagare l'IMU per il 2021 grazie all'azione emendativa della Lega alla Camera dei deputati. Abbiamo tutelato famiglie, imprese, lavoratori autonomi, che non sono in grado di provvedere a tutti gli oneri e gli adempimenti fiscali, che sono stati rinviati caso riteniamo che prima o poi si dovrà parlare seriamente in queste Aule di pace fiscale e di riforma del fisco). Li abbiamo tutelati perché è stato lo Stato a impedire loro di lavorare e ora non può chiedere loro anche di pagare ciò che non sono in grado di pagare. Dobbiamo fare una seria riflessione se oggi ci sono ancora le condizioni in questo Paese per fare impresa, per essere un lavoratore autonomo, per aprire una partita IVA. Il Governo deve dare queste risposte e la Lega insisterà fino alla fine di questo mandato affinché si intervenga seriamente. Noi siamo convinti che sia stato fatto un buon lavoro, un ottimo lavoro. Il decreto-legge in esame, i suoi contenuti, la sua impostazione, i correttivi approvati dalla Camera giustificano pienamente la scelta della Lega di sostenere questo Governo. Se la Lega avesse deciso di stare comodamente all'opposizione senza rischiare, senza assumersi le proprie responsabilità, rimanendo a guardare, a criticare quello che facevano o non facevano le altre forze politiche, molte delle norme utili e necessarie che sono contenute in questo decreto-legge non avrebbero trovato spazio e non avrebbero trovato approvazione da parte delle Aule parlamentari In questa fase così drammatica per il nostro Paese è dovere della Lega garantire il proprio contributo per migliorare, per modificare, per corregge le misure (e anche criticarle quando è necessario) adottate dal Governo. Ci stiamo provando ogni giorno e ci stiamo riuscendo, il provvedimento in discussione ne dà una testimonianza concreta. La maggioranza che sostiene il Governo non è politica, come è evidente a tutti. Nasce in una legislatura in cui nessuno schieramento aveva i numeri per governare autonomamente; le leggi elettorali di Comuni e Regioni garantiscono la governabilità, la legge elettorale delle consultazioni politiche non lo fa. Questa scelta - perché di scelta si tratta - è la vera causa dell'ingovernabilità del nostro Paese e non è una responsabilità della Lega. La pandemia e le sue drammatiche conseguenze non ci consentono di essere inermi spettatori. Questa è la legittima scelta di altri, non la nostra esame ci ripaga pienamente della nostra decisione: aiuta concretamente famiglie, lavoratori, imprese, la nostra collettività, la nostra società a stare in piedi, a reggere e anche ad andare avanti. Senza la Lega al Governo molte delle scelte e delle norme contenute in questo provvedimento non avrebbero trovato spazio, non avrebbero trovato risposta, non sarebbero state approvate. Facciamo però una raccomandazione al Governo che continuiamo a sostenere: non basta stanziare le risorse, bisogna erogarle rapidamente. C'è un ritardo nell'approvazione dei decreti attuativi; chiediamo che ci sia un intervento efficace, solerte, una cabina di regia perché i cittadini non possono aspettare. La nostra parte l'abbiamo fatta, ora sta al Governo stanziare effettivamente le risorse che il Parlamento ha approvato.

Presidente, colleghe e colleghi, componenti del Governo, nell'annunciare il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle alla questione di fiducia posta sul provvedimento in esame, desidero ricordare a tutti i componenti dell'Assemblea che noi siamo qui oggi per fare un altro passo in avanti per vincere questa difficile emergenza. I 45 miliardi del decreto-legge sostegni-*bis* sono un tassello ulteriore del mosaico molto più complesso e corposo di provvedimenti

realizziamo quanto abbiamo già anticipato col precedente decreto-legge sostegni, perché con questo provvedimento sosteniamo con forza le imprese, attenzioniamo i più deboli, supportiamo i lavoratori e le famiglie e aiutiamo anche oltre 1.000 Comuni. che forse dopo un anno non avrebbe nemmeno più senso ribadirlo, però diciamo ancora che è sbagliato e fuorviante pensare alle risorse stanziate in ogni provvedimento per dire se va bene o meno, perché quelle risorse non basteranno mai per le esigenze di tutti; quello che conta, invece, è un percorso che è nato nel marzo 2020 con il decreto-legge cura Italia e del quale poi bisogna tener presente almeno tre elementi. Il primo elemento è quello economico: parliamo di oltre 200 miliardi di euro messi in campo da nove provvedimenti economici nel 2020, dalla legge di bilancio dello scorso anno e dai due decreti-legge sostegni e i 235 miliardi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Fondo nazionale complementare che saranno messi a disposizione da qui ai prossimi sei anni. Infine l'elemento forse più importante: la riapertura graduale delle attività e della filiera economica. Questo, sì, che consentirà di far riprendere finanziariamente il Paese. Oggi dobbiamo ribadire con forza il nostro sostegno alle imprese. In che modo Ci sono 15 miliardi nel provvedimento che sono destinati a contributo a fondo perduto alle imprese e, di questi, 8 miliardi sono automaticamente assegnati ad imprese che già con il precedente provvedimento avevano avuto il contributo a fondo perduto. Se non bastasse questo, vorrei ricordare al collega che mi ha preceduto che lo stesso MoVimento 5 Stelle era concorde nel superare anche la logica del fatturato dopo quella dei codici Ateco. Come l'abbiamo fatto? Si farà riferimento in questo in questo difficile periodo alla perdita di utile avuta dalle imprese, considerando anche i reali costi da esse sostenuti. A questo settore sono dedicati ben 4 miliardi su base opzionale.

perché non solo non ha i genitori o qualcuno che possa dargli una mano, ma perché magari ha avuto un parente da cui ha ereditato una casa e quindi non ha più i requisiti per l'accesso. Come si fa? A queste persone abbiamo pensato quando abbiamo rinnovato di altri quattro mesi il reddito di emergenza.

Per non parlare poi di chi campa di politica da un quarto di secolo - potrei definirli politica dipendenti - che si permette di sputare sulla povera gente, arrivando a dire che il reddito di cittadinanza è il metadone e chi lo percepisce un tossicodipendente. *(Commenti. Applausi)*. Ma vi rendete conto di quello che dite? Cosa sarebbe accaduto in questo periodo se non ci fosse stato il reddito di cittadinanza? Allora noi, oggi più che mai, più di prima, come MoVimento 5 Stelle dobbiamo ribadire che il reddito di cittadinanza si tocca, ma lo si fa per migliorarlo e completarlo.

del decreto-legge sostegni*-bis* superiori a quelli negativi. Per tale ragione stiamo dando fiducia al Governo. Attenzione però, e qui rivolgo un appello al Governo e alle altre forze politiche, affinché nei prossimi provvedimenti si trovi ancora più larga e maggiore condivisione sui temi da trattare.

E qui va il nostro ringraziamento, invece, a tutti i finanzieri e alle Forze dell'ordine per il prezioso lavoro che svolgono quotidianamente, prestando servizio con impegno e dedizione.

Colleghi, è inutile negarlo, siamo politicamente molto diversi e siamo contenti di esserlo. Siamo anche profondamente distanti su temi molto importanti, siamo contenti; tuttavia, vorremmo andare avanti in un percorso di condivisione, seguendo una strada che abbiamo già tracciato, proprio quando abbiamo convertito in legge questo decreto-legge alla Camera. Mi riferisco in particolare all'emendamento votato da tutte le forze politiche - Italia Viva esclusa - che prevede la compensazione dei prezzi per le materie prime nei lavori pubblici. pubblici. Giova a tutti ricordare che la certificazione del credito di imposta, la cessione del credito di imposta e la circolazione "n volte" del credito di imposta introdotta nel maggio 2020 con il superbonus al 110 per cento hanno fatto sì che l'Italia diventasse la prima economia europea a raggiungere i livelli di produzione delle costruzioni addirittura del periodo pre-Covid: l'unica in Europa. *(Applausi)*. Nessun altro è riuscito a raggiungere livelli di produzione delle costruzioni pre-Covid, solo l'Italia. Tanto lavoro però ha generato qualcosa di inaspettato, cioè l'aumento incontrollato di alcuni prezzi dei materiali edili per le costruzioni nei lavori pubblici. Ecco che allora siamo stati bravi, tutti insieme, ad ascoltare le imprese, che ci hanno evidenziato questo problema, e a dare una risposta. Come abbiamo fatto? Abbiamo destinato le somme che sono all'interno dei quadri economici di ogni intervento agli imprevisti e ai ribassi d'asta, inclusi gli accantonamenti non vincolati, per revisionare i prezzi in aumento. Come se non bastasse, abbiamo previsto l'istituzione di un fondo

Dobbiamo lavorare assieme affinché la scadenza del superbonus venga prorogata almeno al 2023 *(Applausi),* in linea con quanto dichiarato dal presidente Draghi nel discorso di insediamento alle Camere. Camere. Soltanto se la scadenza diventa successiva al 2023, possiamo porre termine all'onda speculativa finanziaria generata dall'attuale scadenza, cosicché le imprese possano avere davanti a loro un orizzonte temporale che consenta loro di gestire e organizzare meglio i lavori, generare lavoro in un momento così difficile e soprattutto fare i lavori bene. Signor Presidente, in un momento di così in cui è necessario unire le nostre forze per vincere questa pesante emergenza e far uscire i cittadini italiani e le imprese dalle sofferenze in cui vivono, a nome del MoVimento 5 Stelle esprimo un voto favorevole alla fiducia su questo provvedimento.

Un provvedimento così corposo e importante è arrivato nell'Aula di questo ramo del Parlamento tre giorni fa; è sbarcato in Commissione finanze e in Commissione bilancio con un parere predisposto e letto

politiche - neanche di maggioranza - ha potuto discutere il provvedimento. Si è andati anche oltre, però, questa volta. Addirittura il Parlamento si era espresso in maniera

e sta distruggendo la democrazia in Italia, andando a toccare diritti fondamentali degli individui in assenza di discussione del Senato. L'Alternativa C'è voterà no alla fiducia al Governo Draghi sul decreto la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 2320, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge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 Ricordo che è necessario evitare assembramenti al centro dell'emiciclo. Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale. *(È Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dalla senatrice Pergreffi.

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 2320, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia: | |

Sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 15 con il *question time*.

alle quali risponderanno il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Invito gli oratori ad un rigoroso rispetto dei tempi, considerata la diretta televisiva in corso.

come sappiamo tutti, il Governo ha deciso - a mio parere, giustamente - di prorogare la sospensione dell'esecuzione degli sfratti

stabilisce che gli sfratti esecutivi possano essere eseguiti. Ci sembrava importante confrontarci con il Governo per capire quali misure si possano mettere in campo per fare in modo che questa mole di sfratti,

progressivamente, contingentando i tempi, ma soprattutto perché nessuno resti in strada e che si creino soluzioni per chi viene sfrattato.

dell'interno*. Onorevoli senatori, preliminarmente ricordo che l'articolo 6 del decreto-legge n. 102 del 2013 ha istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli. Lo scorso 8 luglio il Ministero delle infrastrutture, a seguito di intese in Conferenza unificata, ha predisposto per la successiva firma del Ministro dell'economia i decreti di riparto dei fondi di sostegno alle locazioni per un importo di 260 milioni di euro per l'anno 2021. Tale disposizione ha anche previsto il coinvolgimento delle prefetture, attraverso l'adozione di misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto. Anche in relazione alle situazioni di maggiore criticità sul territorio, nella consapevolezza che in molti casi i nuclei familiari oggetto delle procedure esecutive di sfratto si trovano in condizioni di grave disagio economico e sociale, alcune prefetture hanno già attivato tavoli di confronto coinvolgendo i diversi attori istituzionalmente competenti: le Regioni, i Comuni, l'autorità giudiziaria, gli enti di gestione dell'edilizia popolare e le organizzazioni rappresentative dei proprietari e degli inquilini degli immobili. In alcuni casi, si è giunti alla sottoscrizione di un protocollo di intesa con gli interlocutori istituzionali proprio per armonizzare ed integrare gli interventi, in particolare quelli previsti sulla morosità incolpevole sotto i profili della ripartizione delle risorse disponibili, del numero degli alloggi da assegnare in emergenza agli sfrattati, nonché delle procedure da attuare nei confronti delle famiglie colpite da sfratto. Nel quadro delle misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno, con mio decreto del 24 giugno scorso, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, abbiamo ripartito il fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021, previsto dall'articolo 53 del decreto-legge n. 73 del 2021, finalizzato all'adozione da parte dei Comuni di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche in relazione proprio al perdurare dell'emergenza. In conclusione, assicuro che i prefetti, proseguendo nella direzione tracciata fin dall'aprile 2020, a seguito di mia direttiva volta a intercettare i segnali di disagio sociale, ivi compreso quello abitativo, continueranno a svolgere ogni utile iniziativa, anche mediante la sottoscrizione di nuovi protocolli o la rivisitazione di quelli già esistenti, per un'adeguata azione di bilanciamento degli interessi a tutela delle fasce più deboli.

importante. Mi pare che si stiano aprendo i tavoli - la Ministra mi conferma che c'è una direttiva del Governo - per gestire questa fase difficile. Credo che la sensibilità dimostrata meriti un apprezzamento

preso dal sito del Ministero sono più sconfortanti. Per esempio, a Roma al 20 maggio, su un totale di 16.000 di domande ricevute, solo due pratiche sono sono arrivate alla fase conclusiva; a Milano, su 26.000, non più di 400. Secondo me, la scarsa e non entusiasmante applicazione, dovuta - immagino - alle ragioni che ci spiegherà,

ci sarà modo - speriamo che ce lo dica - di sveltire queste pratiche; altrimenti, rischiamo di avere leggi che non si applicano e si accavallano ad altre. Infine, sono contenta che ci sia il Ministro della difesa,

So che alla tabella 7 avete già previsto di portare via tutti gli afghani che ci hanno aiutato e - lo spero bene

A parte loro, se così vanno le cose, cioè se l'Afghanistan torna in mano talebana, e a parte le questioni legate al terrorismo, che vi pregherei di monitorare seriamente, usciranno

preliminarmente va evidenziato che le procedure di emersione hanno incontrato, soprattutto all'inizio, varie difficoltà e tra queste certamente si ascrive la complessità della gara per l'individuazione della società di somministrazione dei lavoratori interinali a supporto degli sportelli unici, l'intreccio delle competenze tra amministrazioni diverse - prefetture, questure, ispettorati del lavoro, INPS nonché l'impossibilità tecnica di gestire la procedura esclusivamente in via telematica. Naturalmente, sull'insieme di tutte queste cause, ha anche gravato l'effetto della pandemia, che ha costretto le strutture periferiche a ridurre gli appuntamenti con gli utenti. Tale situazione contribuisce a spiegare i motivi per i quali alcune importanti realtà provinciali, gravate da un maggior carico di lavoro, tra le quali Milano, Roma e Napoli, registrano tuttora un arretrato nello svolgimento delle istanze, che potrà essere assorbito gradualmente grazie al significativo contributo dei 750 lavoratori interinali, in servizio solo da marzo, a seguito delle procedure di reclutamento espletate dalla società assegnataria dell'appalto. Tale contingente verrà presto incrementato con altre 50 unità. Riguardo ai due distinti procedimenti amministrativi, rispettivamente degli sportelli unici per l'immigrazione presso le prefetture e delle questure, il quadro su base nazionale è il seguente. In relazione al primo procedimento, le domande presentate sono state complessivamente 207.870. Di queste, ad oggi, sono state definite positivamente, all'esito favorevole dell'istruttoria tecnica svolta, 45.173 istanze, con la consegna agli interessati dei moduli per il rilascio dei permessi di soggiorno, di cui 39.292 39.292 per lavoro domestico e assistenza alla persona e 5.881 per lavoro subordinato. Rispetto al totale delle oltre 45.000 istanze, quelle relative al rilascio di permesso per attesa occupazione, vale a dire quelli che non hanno un datore di lavoro, sono state 4.687, di cui 4.439 riferite al lavoro domestico e 248 al lavoro subordinato. Preciso che dello stesso *stock* di domande ne sono state rigettate 4.890, mentre le rinunce sono state 1.331. Dal quadro esposto consegue che gli sportelli unici hanno esitato complessivamente 51.394 pratiche. In relazione alla procedura meno complessa da avviare direttamente presso le questure, informo che rispetto a 11.335 istanze presentate, risultano rilasciati 9.918 titoli di soggiorno.

Ovviamente sono lieta di apprendere che ci sarà un incremento di forze per riuscire a smaltire e ad esaminare tutte le domande. Anche perché, signor Ministro, lei sa meglio di me che queste persone che sono in attesa e hanno anche fatto domanda

Sappiamo che questo strumento ha seguito un percorso particolarmente complesso nella sua messa in servizio. Avevamo lavorato in maniera molto determinata con il suo predecessore, Matteo Salvini, affinché fosse Salvini, affinché fosse messo a disposizione delle nostre Forze dell'ordine e sappiamo che negli scorsi mesi è stata aggiudicata la fornitura di 4.482 pistole a impulso elettrico. Ora si tratta di metterle velocemente a disposizione delle nostre Forze dell'ordine.

*taser* è stato preceduto da una fase sperimentale disposta per motivi precauzionali. Ricordo che il 16 giugno 2020, con mio provvedimento, nelle more della definizione dell'*iter* di adozione n. 359, il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia è stato autorizzato a impiegarla per i compiti istituzionali, a condizione che essa non ecceda le potenzialità offensive delle Forze di polizia. In fase di gara, tuttavia, è stato accertato che mancavano gli *standard* di sicurezza necessari e ciò ha determinato un rallentamento della procedura. In data 7 luglio 2021, dopo tutti gli accertamenti, è stato stipulato il contratto per la fornitura complessiva di 4.482 armi a impulso elettrico, corrispondenti al fabbisogno aggregato di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di finanza. Trascorsi i centoventi giorni previsti dagli atti di gara per la realizzazione della fornitura e all'esito della verifica finale di conformità, le armi con i relativi accessori verranno consegnate alle Forze di polizia. Con riguardo alla valutazione da parte del Governo dell'opportunità di dotare anche gli agenti della Polizia municipale di tale arma, va ricordato che l'articolo 19 del decreto-legge n. 113 consente, a determinate condizioni, ai Comuni capoluoghi di Provincia, nonché a quelli con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, di dotare

di tutela della salute, da adottare a seguito di accordo da sancire in sede di Conferenza unificata. Una bozza delle predette linee generali è stata già sottoposta all'esame della Conferenza unificata in una prima seduta in data 29 ottobre 2019, a a seguito della quale sono state introdotte alcune integrazioni. Più di recente, su richiesta dell'ANCI, l'esame delle citate linee guida è stato rinviato a una prossima riunione tecnica, per verificare con il Ministero della salute la possibilità, per le Regioni e i Comuni, di sottoscrivere specifiche convenzioni nazionale, finalizzate a richiedere personale medico per i moduli formativi in materia sanitaria e di primo soccorso previsti dalle linee guida per il personale delle polizie locali.

tale strumento di difesa (perché di questo bisogna parlare). Dalla sua descrizione deriva comunque un quadro non totalmente soddisfacente, per quanto riguarda i passaggi di burocrazia. È indubbio che il suo impegno e quello del Ministero vadano nella direzione da noi auspicata; è altrettanto vero che bisogna essere molto più determinati nel mettere a disposizione - come dicevo - strumenti di difesa. Badiamo bene: avere a disposizione dei nostri agenti della Polizia, anche della Polizia locale, uno strumento come il *taser* è certamente un deterrente più forte nei confronti di un aggressore, rispetto alla capacità che può avere l'agente della Polizia di intervenire avendo a disposizione la pistola, che è strumento invece atto a offendere e che può portare - come ben sappiamo - anche a tragiche conclusioni. Sapere che invece si ha di fronte un agente della Polizia che ha a disposizione uno strumento che sostanzialmente rende l'aggressore non più in grado grado di aggredire è anche un forte deterrente e consente, in una situazione come quella che stiamo vivendo (anche per quanto riguarda la pandemia), di tenerlo a debita distanza. Se questo strumento sarà velocemente distribuito anche ai nostri Comuni e alle nostre municipalità, saremo ben certi di aver tutelato meglio la sicurezza e

Signor Presidente, signor Ministro, il 2 luglio scorso siamo stati costretti ad abbandonare la base aerea interforze di Al Minhad, negli Emirati Arabi Uniti, operativa dal lontano 2000-2002. Si tratta di una base che è sempre stata necessaria per il supporto delle nostre missioni in Afghanistan (appena conclusa)

generale nello scacchiere mediorientale, e ha sempre garantito il trasporto di personale e di mezzi per i nostri contingenti nazionali impegnati appunto nelle missioni. È quindi, credo, di tutta evidenza la gravità

Si tratta, signor Ministro, di un'area geopolitica di fondamentale importanza, essendo la base emiratina, come saprà, l'unica in grado di supportare le missioni italiane nell'area. Aggiungiamo anche che questa determinazione prepotente del Governo emiratino appare come una ritorsione, a seguito di alcune decisioni del Governo *pro tempore* Conte II, ovvero quelle di revocare talune commesse e forniture di carattere militare. Non entro in questo argomento che non compete la Difesa, ma è evidente - e questo invece riguarda anch'essa - che c'è una situazione di crisi e di tensione diplomatica e politica tra il nostro Paese e gli Emirati Arabi. Questo potrebbe anche compromettere la nostra partecipazione col pattugliamento marittimo nello stretto di Ormuz, che ha bisogno di quell'area come base. Fratelli d'Italia chiede di sapere fondamentalmente tre questioni. Intanto, vorremmo sapere se non ritenga che questa vicenda abbia danneggiato gravemente l'immagine dell'Italia a livello internazionale.

terzo e ultimo punto, non irrilevante, riguarda la sorte e il destino degli strumenti e dei materiali appartenenti alla Difesa italiana e se si ipotizza in questo un danno erariale per lo Stato italiano, in quanto difficilmente potranno essere recuperati.

in merito al quesito posto dall'interrogante, come noto, le autorità emiratine hanno recentemente comunicato, tramite l'addetto militare di Abu Dhabi, la volontà di non estendere il Memorandum of understanding (MOU) tra il comando generale delle Forze armate degli Emirati Arabi Uniti e la Difesa italiana. Al riguardo, il comando operativo di vertice interforze ha disposto l'immediata esecuzione del rischieramento di tutto il personale, degli aerei e del materiale presente nella Forward logistic air base di Al Minhad, riposizionando parte del dispositivo in Kuwait. In particolare, dei 142 militari in forza alla base, 79 sono stati rimpatriati, 40 sono stati rischierati in Kuwait, per garantire la capacità di evacuazione sanitaria di urgenza e il trasporto tattico, mentre 23 sono rimasti in forza all'ufficio coordinamento transizione, dislocato a Dubai con funzioni di nucleo stralcio. Nello specifico, quest'ufficio sta assolvendo i compiti di chiusura delle pendenze di natura amministrativo contabile, ivi comprese le procedure per il rilascio delle aree in uso al contingente nazionale presso l'aeroporto di Al Minhad. Nonostante il limitato preavviso ricevuto delle autorità emiratine, è stato tecnicamente possibile rimpatriare e movimentare materiali sensibili, attrezzature, mezzi e velivoli. In particolare, sono stati riposizionati, presso il sedime di Al Salem in Kuwait, automezzi, gruppi elettrogeni, sistemi di comunicazione, armamento, materiale sanitario, parti di ricambio dei veicoli e equipaggiamenti della linea volo e per le esigenze di manutenzione. In merito all'*hangar* manutenzione, ai moduli prefabbricati, agli alloggi, alla mensa e alle aree ricreative, nonché agli arredi, è tuttora in atto, da parte del citato nucleo stralcio, la definizione delle procedure tecnico-amministrative per la corretta individuazione della destinazione d'uso, non essendone stato tecnicamente possibile lo smontaggio e il rimpatrio in considerazione delle ridotte tempistiche disponibili. Le conseguenze della decisione emiratina sull'attività di rientro del contingente italiano dall'Afghanistan sono state pienamente superate, grazie alla capacità del comando operativo di vertice interforze di adattare il piano di ripiegamento alla nuova situazione, utilizzando strutture alternative senza subire ritardi. Come ho già avuto modo di dire nel corso della mia audizione lo scorso 7 luglio in Commissione quadrangolare esteri e difesa, la Difesa guarda con attenzione alle azioni diplomatiche in corso, per la ripresa del dialogo e la ricomposizione di positive relazioni con quello che rimane un *partner* importante per il nostro Paese. Tali valutazioni e tale attenzione sono accompagnate da impressioni positive anche in relazione al dialogo che ho avuto con il mio collega emiratino. Ciò detto, non ritengo che questa vicenda abbia scalfito in alcun modo l'immagine delle Forze armate italiane, anche per via della grande credibilità, unanimemente riconosciuta, alle nostre donne e ai nostri uomini in uniforme impegnati nel loro apprezzatissimo servizio in Italia e all'estero.

per quello che abbiamo sentito, molto lo sapevamo già ed è stato anche oggetto di alcune nostre interrogazioni, rimaste peraltro senza risposta. Soprattutto, però, ci delude quello che non abbiamo sentito, ovvero il fatto che il Governo non abbia mai speso una parola di apprezzamento per il contingente che, in meno di due settimane, ha dovuto smantellare un'intera base come quella di Al Minhad, oltre a difendere e salvare i nostri materiali.

stupisce ascoltare che questo non abbia leso la nostra immagine. Signor Ministro, mi scusi, non è colpa sua, ma l'Italia ha subito un sonoro ceffone da questa storia e perché è una ritorsione e perché è una prepotenza - e non mi pare di aver letto, né sentito una voce che abbia difeso il prestigio della Nazione, l'autorevolezza delle missioni internazionali e l'interesse nazionale. Mi pare che ci sia la volontà di stendere un manto di silenzio, perché abbiamo perso, non solo la base, ma, me lo lasci dire, anche la faccia. È questo che noi abbiamo perso a livello internazionale, signor

dopo certe vicende, in un contesto ben diverso, in un'Europa dove i valori della pace e della convivenza si affermano e credo sia doveroso ricordare in maniera adeguata questo evento. In occasione di un anniversario così importante in termini morali ed educativi, come sottolineato anche dal Presidente della Repubblica nel discorso di fine anno e come ribadito più volte dallo stesso Ministro della difesa nel corso dell'intervento sulle linee programmatiche del Ministero, la memoria e la consapevolezza della nostra identità nazionale ci aiutano a costruire il futuro.

dunque, in conclusione, di conoscere se e quali iniziative si stanno predisponendo per la commemorazione di questo evento, anche al fine di non disperdere il significato della memoria storica, quale patrimonio culturale collettivo, da trasmettere e diffondere, anche tra i giovani, unitamente agli indefettibili obiettivi di educazione, formazione e partecipazione. Quindi, signor Ministro, vorremmo che anche il Senato potesse associarsi a questi momenti di celebrazione e conoscere le scadenze previste.

di rispondere a tale interrogazione, condividendo in pieno le motivazioni poste alla base del meritorio indirizzo espresso in merito dal Parlamento e appena ricordato dal senatore interrogante. Sui simboli e sui loro significati non ci si può dividere; è anzi doveroso travasarne la forza unificatrice alle giovani generazioni, perché il messaggio che ci donano integra, rafforza e si armonizza con gli obiettivi di educazione, formazione e partecipazione, che possono rendere proprio i giovani gli attori protagonisti del ricordo di un passato nobile che, loro tramite, diviene futuro. Nel merito dei quesiti posti, sono numerose le iniziative in cui la Difesa svolge un ruolo da protagonista o da agenzia di coordinamento e supporto, per consentire un quadro di pieno decoro agli eventi commemorativi.

che coinvolge le amministrazioni comunali per il conferimento della cittadinanza onoraria al Milite ignoto. A supporto sono impegnati il Commissariato generale per le onoranze ai caduti, nonché lo Stato maggiore della difesa e i comandi militari territoriali. Sono lieto di condividere con voi il raggiungimento delle prime 2.000 adesioni da parte dei Comuni italiani. L'apertura delle celebrazioni si è già avuta lo scorso 1° giugno presso il Salone delle bandiere dell'Altare della Patria, con un evento che ha visto una partecipazione qualificata, arricchita da intellettuali, giornalisti ed attori, oltre che rappresentanti istituzionali. Nel mese di giugno, una vettura militare storica, personalizzata con i simboli dell'anniversario, è stata impegnata nella Mille Miglia, la corsa più bella del mondo, portando il simbolo del centenario nelle strade d'Italia, in un contesto prestigioso che ben gli si addice. A sottolineare il profondo valore culturale della ricorrenza e l'obiettivo di coinvolgere i nostri concittadini più giovani, lo Stato maggiore della difesa sta organizzando, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, un convegno storico sulla figura del Milite ignoto, che sarà condotto in modalità *streaming* e utilizzando la realtà virtuale per una rappresentazione realistica dei contesti in cui queste vicende ebbero luogo. Inoltre, all'apertura del prossimo anno scolastico verrà indetto un concorso sul tema, che coinvolgerà tutte le scuole di ogni ordine e grado. Allo scopo di rendere idealmente omaggio ai milioni di soldati, che dalle più remote località natie raggiunsero i fronti di guerra, il prossimo 28 ottobre partirà dalla stazione ferroviaria di Aquileia il treno della memoria, che, ripercorrendo le tappe storiche del viaggio della traslazione, giungerà a Roma conducendo idealmente le spoglie del caduto. Questa fase culminerà con la solenne manifestazione del 4 novembre, presso l'Altare della Patria, alla presenza delle più alte cariche istituzionali. Questo viaggio, per il quale si deve gratitudine alle Ferrovie dello Stato e alla loro Fondazione, proseguirà verso il Sud Italia, ma è toccato prima dal convoglio, per quello che vuole essere un abbraccio unificatore all'intero Paese. I dettagli di questa attività, della speciale mostra che verrà realizzata a novembre al Sacrario delle bandiere,

Numerose sono anche le iniziative collaterali per una serie importante di eventi che, con la necessaria attenzione alle condizioni sanitarie e il fondamentale supporto istituzionale, suggelleranno in modo indelebile i cento anni di uno dei simboli più puri e sorprendentemente moderni sui quali poggia il nostro concetto di unità nazionale.

del viaggio del treno che da Aquileia ripercorrerà le tappe della traslazione del corpo del Milite ignoto all'Altare della Patria - mi è venuta un'idea. Ho visto qualche volta in televisione le immagini di quel viaggio; a volte capitano a tarda notte, su Rai Storia, su canali importanti. Colgo l'occasione per invitare anche lei, come membro del Governo,

di ulteriore consolidamento del sentimento di appartenenza alla Nazione. Non è un caso, poi, che il bollettino della vittoria sia riproposto in tante sedi: anche noi lo abbiamo in un luogo di passaggio tra i palazzi del Senato, nel cortile che porta verso il palazzo delle Commissioni, a dimostrazione che in tutti i luoghi pubblici quell'evento ha segnato e scandito l'unità nazionale. Pertanto, l'onore al Milite ignoto sarà un momento importante di riflessione, anche per le prospettive odierne e future di un'Europa che non dimentichi la storia e l'identità delle singole Nazioni.

signor ministro Orlando, propongo questa interrogazione perché un grave fatto di cronaca ha riportato alla nostra giusta attenzione il tema della molestia sui luoghi di lavoro e per sapere quale programma abbia il Governo, lei e in particolare il Ministero che guida, per rendere i posti di lavoro liberi dalle discriminazioni, dal *mobbing*, dallo *straining*; in una parola, per rendere il lavoro realmente dignitoso e i lavoratori liberi di esprimere il meglio di sé sui posti di lavoro.

però noi riteniamo che ancora manchino gli strumenti attuativi e delle leggi di dettaglio che rendano realmente operativi questi validissimi principi che il nostro ordinamento si è dato. Il fatto a cui mi riferisco è successo il 4 marzo scorso in Trentino, quando una giovane ginecologa è scomparsa; le indagini sono ancora in corso, così come le ricerche. Ciò che è noto è che il giorno precedente, il 3 marzo, la dottoressa Pedri Sara (questo è il suo nome) ha rassegnato le proprie dimissioni dell'azienda sanitaria e ha raccontato ai propri familiari di essersi tolta un peso con questo gesto. Tutto il resto, tutto l'altro che sappiamo lo conosciamo grazie al meritorio lavoro dei giornalisti, della stampa che ha acceso un faro sulla vicenda e sul tema delle molestie sul luogo di lavoro. Raccontano di turni massacranti, di abusi di potere, di minacce continue e per questo il 23 giugno scorso ho interrogato il Ministro della salute, affinché potesse inviare degli ispettori all'ospedale di Trento, in particolare nel reparto di ginecologia. Il ministro Speranza ha prontamente inviato gli ispettori e stiamo attendendo di leggere la loro relazione. Ministro, questo fatto deve porre alla nostra attenzione un tema: anche in realtà sanitarie di grande eccellenza, che sembrano primeggiare in Italia nelle classifiche per la qualità delle prestazioni, per la competenza dei medici e degli operatori, possono accadere gravi problemi di ordine organizzativo e di qualità delle condizioni di lavoro. Mi pare dunque urgente

Signor Presidente, desidero davvero ringraziare gli onorevoli interroganti per aver voluto, con questo atto di sindacato ispettivo, mantenere alta l'attenzione su un episodio drammatico che ha molto colpito l'opinione pubblica. Al riguardo intendo dare atto a tutte le istituzioni di essersi immediatamente attivate per fare chiarezza su quanto avvenuto e sulle eventuali responsabilità. La vicenda di Sara Pedri impone una riflessione generale che deve essere compiuta in un'ottica di sistema. Il fenomeno della violenza nei luoghi di lavoro pone in rilievo diritti e principi di rango costituzionale e diritti inviolabili dell'uomo anche nell'ambito delle formazioni sociali: il diritto alla salute e all'integrità psicofisica, il rispetto della libertà e della dignità umana nell'ambito dell'iniziativa economica. Inoltre, è ormai unanimemente riconosciuto che tali fenomeni, oltre alle sofferenze e al disagio a carico della vittima e del suo nucleo familiare, generano ingenti costi diretti e indiretti che si traducono in criticità anche nell'ambito degli ambienti lavorativi. Per tale motivo è stato dato un forte impulso ad intervenire sul piano normativo con l'entrata in vigore della legge n. 4 del 2021, di ratifica della convenzione ILO n. 190, al fine di introdurre una tutela adeguata del nostro ordinamento e in aderenza agli standard di prevenzione e protezione contenuti nella disciplina internazionale. A tale riguardo credo che sia importante segnalare che la convenzione stabilisce, tra gli altri, l'obbligo di adottare misure volte a conferire poteri più incisivi agli ispettorati del lavoro e ad attribuire e ad attribuire il potere di adottare, ove necessario, misure immediatamente esecutive. Con riferimento alla tutela del lavoratore e ad eventuali ritorsioni in ambito lavorativo, desidero segnalare che stiamo procedendo, congiuntamente con il Ministero della giustizia e con altre Amministrazioni coinvolte, al recepimento della direttiva n. 1937 del 2019, con il preciso scopo di assicurare un'adeguata tutela ai lavoratori che decidono di denunciare irregolarità e illeciti di cui siano venuti a conoscenza nel proprio luogo di lavoro. Condivido quindi l'opportunità di valutare l'iniziativa legislativa *ad hoc*, nel senso auspicato dagli interroganti, che integri le forme di tutela finora garantite in massima parte per via giurisprudenziale, al fine di uniformare la definizione della fattispecie del *mobbing*, ampliare la conoscenza del fenomeno, anche in relazione agli aspetti di organizzazione del lavoro, potenziare le politiche di prevenzione ed introdurre misure più efficaci di contrasto. Si tratta di interventi che necessitano comunque di una strategia comune in materia di tutela di diritti, di salute e di sicurezza del lavoro. Occorre altresì potenziare percorsi già avviati con le parti sociali e con il consigliere di parità per l'attuazione degli impegni assunti nel contesto dell'accordo siglato nel 2016 tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL, il quale recepisce l'accordo quadro sulle molestie e la violenza sui luoghi di lavoro raggiunto a livello europeo. Le parti sociali rappresentano infatti anche in quest'ambito uno snodo fondamentale per favorire la realizzazione di cambiamenti positivi sul posto di lavoro, per proteggere i lavoratori e adottare azioni e progetti che possano prevenire le condizioni generatrici di violenza. Sono pertanto disponibile ad attivare un percorso di confronto tecnico anche con le altre amministrazioni interessate, a partire da salute e giustizia, e ovviamente offrire piena disponibilità al confronto anche rispetto ad eventuali iniziative legislative cui il Parlamento intenda dare corso.

in questa replica di imprimerle il senso di urgenza dettato da questo caso specifico, che forse avrebbe potuto essere evitato con delle misure più puntuali di difesa e di tutela dei lavoratori e per tutti gli altri lavoratori che hanno sofferto e che stanno soffrendo.

imprime dei principi generali alti che però necessitano di misure attuative per essere riempiti di contenuto. Mi riferisco, ad esempio, al principio generale della tutela dei testimoni; è difficile provare una violenza o il *mobbing.* È altresì difficile avere dei testimoni a supporto. Per questo è importante non solo affermare il principio, ma anche dotare il nostro ordinamento di strumenti che definiscano la situazione, che siano per esempio nulli licenziamenti, demansionamenti e trasferimenti. È importante dare la necessità e quantificare i risarcimenti, non solo quelli patrimoniali, ma anche i risarcimenti dissuasivi. Per questo, Ministro, ci sono dei disegni di legge studiati e scritti bene che il Parlamento propone all'attenzione del Governo, soprattutto a tutela di tutti

Ad oggi purtroppo il lavoro dell'operatore socio-sanitario non è riconosciuto come gravoso e, di conseguenza, gli OSS non possono accedere al prepensionamento in presenza degli opportuni requisiti di legge. Infatti il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5 febbraio 2018, che ha provveduto alla specificazione delle professioni individuate alla lettera *f),* dell'allegato B, della legge n. 205 del 2017, alla voce addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza ha inserito esclusivamente il codice Istat 5.4.4.3. Questo ricomprende al suo interno la professione di operatore socioassistenziale, cosiddetto OSA, ma non quella affine, in quanto a funzioni e a gravosità delle mansioni, dell'operatore socio-sanitario, indicata invece con il codice Istat 5.3.1.1.0. Quindi l'OSA può accedere al prepensionamento per aver svolto lavoro gravoso in presenza dei requisiti di legge; l'OSS, invece, pur in presenza dei requisiti di legge, non Sottolineo che le due professioni differiscono esclusivamente per la maggior formazione e responsabilità che caratterizza la figura dell'operatore socio-sanitario. Alcuni datori di lavoro per superare il problema hanno squalificato i dipendenti da OSS ad OSA, strada sicuramente pericolosa, che non rende di certo giustizia degli anni già trascorsi nello svolgimento del lavoro di OSS. È quindi necessario superare questa ingiustificata disparità di trattamento tra professioni molto simili. Alla luce di quanto detto, Ministro, le chiediamo anzitutto anzitutto se sia a conoscenza di quanto esposto, nonché se ne sia a conoscenza la commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, istituita dalla legge n. 160 del 2019, e quali valutazioni stiate facendo sia lei che la commissione in parola;

gli onorevoli interroganti pongono il tema della revisione, della classificazione e specificazione delle categorie lavorative gravose, ai sensi del decreto interministeriale del 5 febbraio 2018, con particolare riferimento al riconoscimento in quanto a funzioni e a gravosità delle mansioni dell'operatore socio-sanitario. Si tratta di una professionalità che svolge - nell'ambito delle proprie competenze - importanti attività di assistenza, cura e prevenzione. Peraltro, a seguito dell'approvazione di un emendamento da parte della Camera dei deputati in sede di conversione del decreto-legge sostegni-*bis*, è stato riconosciuto l'inserimento della professione degli OSS nel ruolo socio-sanitario. In via generale non vi è dubbio che occorre procedere a un aggiornamento della classificazione delle occupazioni gravose, al fine di considerare le specificità delle condizioni attuali di vita e di lavoro e garantire maggiore equità nel sistema dei benefici pensionistici. Non tutte le mansioni gravose e usuranti sono infatti oggi adeguatamente riconosciute e tutelate. Per questo, ho ritenuto prioritario attivare la commissione tecnica, incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, istituita lo scorso novembre. Il 5 maggio scorso è tornata a riunirsi, dopo la modifica della sua composizione conseguente alla nascita del nuovo Governo. Compito della commissione è valutare l'impatto sull'aspettativa di vita di talune condizioni di lavoro per meglio analizzare e studiare le risposte previdenziali più adatte a specifiche categorie professionali. I lavori della commissione sono ancora in corso, essendo stato prorogato al 31 dicembre 2021 - ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto-legge n. 183 del 2020 - il termine previsto per la conclusione dei lavori. Riguardo all'attività della commissione, si evidenzia comunque che, grazie al contributo tecnico-scientifico, offerto, tra gli altri, da INAIL, Istat e INPS, è attualmente in corso una puntuale ricognizione sia delle categorie per le quali sono già oggi riconosciuti i benefici pensionistici riservati alle occupazioni gravose sia nei confronti di altre che potrebbero essere ad esse assimilate in quanto caratterizzate da indici di faticosità e rischiosità particolarmente elevati. In tale prospettiva di studio sono esaminati anche i profili finanziari connessi alla predisposizione di eventuali interventi normativi di riordino della materia, con ridefinizione pertanto delle categorie lavorative considerate gravose. Il lavoro della commissione rappresenta quindi un'occasione molto importante per procedere a un aggiornamento del quadro delle gravosità delle attività lavorative e arrivare a un nuovo sistema che risponda alle esigenze dei lavoratori e delle lavoratrici. In tale ambito potrà essere certamente sottoposta a valutazione la richiesta degli onorevoli interroganti. I presupposti sui quali si sta muovendo la commissione incoraggiano a pensare che tutta una serie di attività che che rientrano negli indici indicati possano essere prese in considerazione. Attendiamo, però, l'esito di questo tipo di analisi, sulla base del quale sarò in grado di dare una risposta compiuta.

Signor Presidente, la vittoria della nazionale di calcio agli Europei, le campionesse del mondo della pallavolo *under* 21, il successo di Berrettini sono motivo di orgoglio e felicità per tutti noi. In questo momento così difficile, lo sport, il colore azzurro,

nazionale e culturale. Per questo, vorrei ringraziare tutti gli atleti e le atlete che parteciperanno alle Olimpiadi di Tokyo e permettetemi e permettetemi di rivolgere un augurio particolare ai quattro atleti della mia città, Fiumicino. Questi atleti sono l'orgoglio di un Comune come tanti, che ha sofferto per questa pandemia, a causa della crisi del settore turistico,

che partecipano ad un evento sportivo così importante è un onore per la nostra città. Vorrei fare i loro nomi: Daniele Lupo, Giordana Sorrentino - una donna - per il

La decisione se riaprirle o meno è un tema che le sta portando all'attenzione pubblica. In realtà, dietro questo settore c'è una generazione economica molto importante, soprattutto degli imprenditori che pagano tasse, che hanno dipendenti, che stanno facendo grandissimi investimenti. Cito Cito un imprenditore riminese, Enrico Galli, che nel febbraio 2020 ha acquistato una delle discoteche più importanti d'Italia e a fronte di un investimento molto alto, in 17 mesi ha aperto solo per qualche serata. È un momento molto difficile per questo settore. Il ministro Garavaglia ha dato una grande disponibilità per discutere il tema di una riapertura, in questo momento, ordinata, coordinata e precisa. Attualmente, ogni angolo delle nostre città sta diventando una discoteca assolutamente fuori controllo: ci sono feste da tutte le parti, notevoli problemi di ordine pubblico che i locali in realtà possono gestire. Ci vuole assolutamente molta prudenza in questo momento, quindi ringrazio il Ministro per la disponibilità il lavoro che sta facendo con il comitato tecnico-scientifico per poter riaprire con delle linee guida corrette, perché è assolutamente importante mantenere la salute pubblica al centro di ogni dibattito. Auspico che questo settore, che è stato colpito in maniera molto forte dalla pandemia, possa avere ristori e aiuti sufficienti. In realtà, tale settore viene sempre collegato ai giovani, ma tocca tutte le generazioni in maniera trasversale.

del FUS e di ammortizzare l'IVA come tutti gli altri settori culturali e come avviene in tutti gli altri Paesi d'Europa. Bisogna soprattutto abolire la tassa sull'intrattenimento e intervenire sull'articolo 100,

alla macchina della giustizia civile. Parlo di un corpo di norme molto importante che interessa quasi tutti gli istituti della procedura civile e, tra questi, anche l'esecuzione civile. Abbiamo letto con amarezza quanto riportato a pagina 57 del PNRR,

questa legislatura. Riteniamo tali norme di buonsenso perché vanno a contemperare gli interessi sia del creditore che del debitore, un compito molto difficile in un campo minato, molto delicato come quello delle esecuzioni immobiliari.

dispongono una serie di misure che intervengono sulle procedure esecutive come, ad esempio, quelle che riguardano le aste giudiziarie, che consentono all'esecutato, la cui abitazione è sottoposta a vendita agli incanti, di continuare a vivere insieme alla famiglia nella propria abitazione anche dopo l'aggiudicazione e fino a un termine congruo - penso sia di sessanta giorni - che consente all'esecutato di cercare

Un mancato controllo della situazione potrebbe determinare una condizione di *caos* come, ad esempio, l'aumento dei suicidi, l'aumento nelle periferie di vere e proprie *bidonville*, di vivai per la criminalità organizzata.

Queste persone, invece, contano su di noi e, quindi, faccio un appello a tutto il Parlamento e al centrosinistra di non votare norme che vadano ad abrogare la normativa attuale. Faccio un appello a Fratelli d'Italia, che continua a essere folgorata sulla via di Damasco, non soltanto perché ritiri questi emendamenti, ma anche perché voti contro quelli che vanno in questo senso.